L ’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 7 ottobre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute: «Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»

(M5S). Signor Presidente, desidero portare all’attenzione dell’Assemblea e dei colleghi l’ennesimo balzello a danno dei cittadini, già tartassati, in una fase economica drammatica come questa per le famiglie, da parte del sistema nazionale per i pagamenti PagoPA (pubblica amministrazione), realizzato dall’Agenzia per l’Italia digitale, che avrebbe il dovere di rendere la vita più facile per il consumatore, invece di continuare a vessarlo. Sollecito contestualmente la risposta all’interrogazione 4-04167. Con tale sistema unico, i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione (come tasse, multe, bolli, visite ASL, utenze, mense scolastiche, rete universitaria e molto altro) non vengono convogliati in un unico sito, ma districati tra diversi canali telematici, siti e app dei tanti enti pubblici, Comuni, Regioni e università, sui quali poter pagare oppure chiedere all’ente un avviso di pagamento, cioè un bollettino cartaceo, da pagare attraverso altri canali, quali sportelli fisici, ATM, siti web, app di banca e così via. Digitalizzare i processi comporta la possibilità di fare tutto on line, senza uscire di casa e senza fare code, mentre in realtà i cittadini devono ancora districarsi, come detto, tra bollettini cartacei.

mentre in precedenza alcuni pagamenti domiciliati in banca erano gratuiti, adesso noi abbiamo un balzello da 2,50 a 2,85 euro. Il codice del consumo le norme di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento vietano l’applicazione di commissioni sui pagamenti elettronici. Chi compra on line un biglietto aereo o fa la spesa sul sito del supermercato non deve pagare una commissione, in quanto ha effettuato il pagamento con carta di credito o altra modalità digitale e questo vale anche per i pagamenti

certi della domiciliazione bancaria (e qui rivolgo un appello a tutti, anche ai senatori), potrebbero per errore ignorare l’avviso di pagamento, diventando così morosi, visto che non c’è mai stata una campagna capillare di informazione, configurando persino un danno erariale. Concludo, signor Presidente e la ringrazio. Pagare quella che agli occhi dei cittadini è considerata una tassa sulla tassa rappresenta sempre un’ingiustizia, tanto più che a favore dei negozi e dei professionisti…